la giustizia*. Con riferimento all'interrogazione del senatore Zanettin, voglio precisare che l'istituzione o la soppressione di uffici giudiziari, al di fuori dei casi tassativamente previsti (che riguardano soltanto le sezioni distaccate di tribunale e gli uffici del giudice di pace), è disposta non con atto amministrativo ma con un atto avente forza di legge e, pertanto, può essere effettuata esclusivamente a seguito di una iniziativa legislativa, che allo stato non c'è. Si rassicura comunque il senatore interrogante che non soltanto - come ho detto - non è in corso alcuna specifica iniziativa legislativa in ordine alla geografia giudiziaria e quindi neppure per quanto riguarda il tribunale interessato, Bassano del Grappa, ma, più in generale, valutate approfonditamente le attuali necessità organizzative degli uffici giudiziari e le possibili soluzioni, non sussiste alcuna intenzione di variare la "geografia giudiziaria" delle sedi di tribunale. Quando il Ministro, nell'audizione sia alla Camera che al Senato, fece cenno alla revisione delle disposizioni giudiziarie, nel senso di eventualmente accorpare sezioni distaccate ad altri tribunali, non indicò alcun tribunale da sopprimere nè tampoco il tribunale di Bassano del Grappa. Quindi, gli eventuali ritocchi, sempre da compiere con atti amministrativi specifici, possono riguardare allo stato soltanto sezioni distaccate e non i tribunali. Per essi confermo che non c'è alcuna iniziativa legislativa al riguardo. Quindi posso rassicurare pienamente il senatore Zanettin che nulla allo stato né in prospettiva di prossimo futuro o di futuro può riguardare il tribunale di Bassano del Grappa.

per queste rassicurazioni che ha voluto fornire alla comunità locale di Bassano del Grappa, rimasta molto allarmata quando erano state pubblicate delle indiscrezioni di stampa, in particolare su "Il Sole 24 Ore", che paventavano appunto la chiusura del tribunale di Bassano del Grappa.

tra organici della magistratura, personale di cancelleria e numero di abitanti, nonché un'area che, come lei ben sa, Sottosegretario, è molto sviluppata dal punto di vista economico e, quindi, necessita di pronte risposte da parte della giustizia. Quindi non posso che prendere atto con favore e con piacere della sua risposta rassicurante per tutta la comunità locale. Non posso, anche in questa occasione, sottacere comunque il grave disagio che, in particolare, il Veneto sta soffrendo per quanto riguarda il rapporto tra magistrati disponibili e carichi pendenti. Approfitto di questa occasione per sollecitare il Ministero della giustizia a rispondere ad altre mie interrogazioni che riguardano altri uffici giudiziari particolarmente compromessi in questo momento nel rapporto appunto tra carichi pendenti e possibilità di esito positivo dei carichi stessi, in particolare per quanto riguarda gli uffici giudiziari del tribunale di Vicenza. Quindi le raccomando grande attenzione per questi uffici giudiziari che hanno bisogno di interventi significativi da parte del Ministero nell'interesse precipuo dei cittadini che attendono giustizia.

In particolare la senatrice Boccia rappresenta che, durante un incontro con i detenuti in occasione di una sua visita alla casa circondariale di Nuoro in data 1 novembre 2006, il Musumeci, anche alla presenza del direttore dell'istituto di pena, riferì di un episodio di percosse avvenuto nel carcere da parte di un ufficiale o un comandante dei Carabinieri in danno di altro detenuto. Gli interroganti lamentano che a causa di tali dichiarazioni il Musumeci punito, ma che la sua condotta non integra gli estremi di una infrazione disciplinare e quindi non doveva essere sanzionata. Le notizie acquisite presso la direzione della casa circondariale di Nuoro a seguito dell'interpellanza sono le seguenti. Il Musumeci, condannato in via definitiva alla pena dell'ergastolo, si trova ristretto in regime detentivo speciale ai sensi dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, regime adottato in situazioni di emergenza. In data 13 luglio 2006 si è fatto promotore ed ha diffuso anche ad organi di stampa una lettera aperta in cui si preannunciavano manifestazioni di protesta a causa del "pestaggio" posto in essere nei confronti del detenuto di cittadinanza albanese Hiseny Hamit. Per la diffusione di tali notizie la procura della Repubblica di Nuoro, a seguito di indagini, ha aperto un procedimento penale a carico del Musumeci e di altri 14 detenuti, ipotizzando i reati di calunnia, diffamazione e diffusione di notizie false. In questa circostanza è stata contestata al predetto l'infrazione disciplinare prevista dall'articolo 77 del regolamento penitenziario, e cioè "promozione di disordini e sommosse", e la conseguente sanzione dell'esclusione dalle attività in comune per sette giorni. Per quanto concerne la vicenda del cittadino Hamit, la direzione del carcere ha chiarito che, in data 8 luglio 2006, al fine di frenare una violenta reazione del detenuto che tentava di sottrarsi ad una perquisizione personale, si è reso necessario l'intervento di agenti di Polizia penitenziaria (non dei Carabinieri). Per tale fatto l'Hamit è stato denunciato alla procura della Repubblica di Nuoro, le indagini si sono concluse e il predetto risulta imputato dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Allorché, in data 1° novembre 2006, il Musumeci, volendo riaccendere la questione, ha riferito la vicenda Hamit alla senatrice Boccia, riproponendo le accuse nei medesimi termini nonostante le indagini dei magistrati, la direzione del carcere ha ritenuto di contestargli nuovamente l'infrazione prevista dall'articolo 77 e di irrogare la sanzione dell'esclusione dalle attività comuni per dieci giorni. Al fine di chiarire ulteriormente l'accaduto, sono state richieste informazioni anche in merito a tale cittadino albanese, il quale, all'epoca del fatto, è risultato essere detenuto in regime di elevato indice di vigilanza, per espiare una pena di oltre sei anni a seguito di una condanna per spaccio di sostanze stupefacenti, falsità materiale e ricettazione. Per essere più preciso nei confronti degli interroganti, occorre preliminarmente rilevare che il Musumeci sicuramente non ha assistito all'episodio concernente le percosse e pertanto egli ha divulgato la notizia senza vera cognizione di causa; per tale motivo ha anche riferito che un comandante dei Carabinieri avrebbe partecipato al presunto pestaggio, circostanza impossibile, in quanto l'Hamit si trovava già in espiazione pena e quindi l'unica polizia che poteva intervenire all'interno dell'istituto carcerario era quella penitenziaria. E l'accaduto, infatti, è stato in realtà diversamente ricostruito dai magistrati, i quali hanno addirittura rinviato a giudizio l'Hamit. secondo luogo, la condotta del Musumeci, che ha sollecitato reiteratamente le proteste dei detenuti con il pretesto del presunto pestaggio, ha sicuramente generato preoccupazione per l'ordine e la sicurezza dell'istituto ed è per tale motivo che la direzione ha adottato le misure in questione. La sanzione disciplinare irrogata, debitamente contestata all'interessato secondo le norme dell'ordinamento penitenziario, risulta, peraltro, la più lieve tra quelle previste dall'articolo 39 del medesimo penitenziario e quindi appare adeguata al fatto ed al comportamento del Musumeci, il quale non ha ritenuto neppure di proporre reclamo al magistrato di sorveglianza o agli altri organi competenti, come avrebbe potuto.

il contesto di alcune di queste situazioni è abbastanza difficile. Di conseguenza, il Ministero conosce bene la drammaticità di tale realtà, soprattutto in quel carcere. In questa situazione

di una situazione più generale che veniva denunciata dai detenuti che partecipavano al colloquio: la mancanza, cioè, di qualsiasi forma di dialogo, di ascolto e di rapporto

Spa, principale produttore sud europeo di carte grafiche prevalentemente patinate per la stampa di cataloghi, riviste, stampati commerciali e libri. A seguito della perdita avvenuta nel 1999 del cliente principale dello stabilimento, cioè della SEAT Pagine Gialle, il Gruppo ha provveduto ad una riconversione specializzandosi sempre più nella produzione di carta riciclata, fino a raggiungere la certificazione ECOLABEL che, come si sa, qualifica le aziende dal punto di vista del ciclo produttivo rispettoso dell'ambiente. A causa di ulteriori difficoltà di mercato di questo prodotto e dei costi crescenti (soprattutto di energia), comuni peraltro a tutto il comparto cartario nazionale, Spa hanno manifestato la propria ferma volontà di cessare la produzione nello stabilimento di Lama di Reno. Il gruppo si è dichiarato disponibile però a cedere lo stabilimento a un soggetto imprenditoriale, anche concorrente, purché intenzionato a proseguire l'attività produttiva e, quindi, a garantire i livelli occupazionali. Tale volontà è stata ribadita più volte, nonostante nei mesi scorsi fosse stato avviato il confronto sul progetto «La filiera delle cartiere», presentato opportunamente dalle istituzioni locali in collaborazione con le altre aziende del settore presenti nella zona, insieme all'università e con la diretta partecipazione delle organizzazioni sindacali. La decisione dell'azienda di dismettere lo stabilimento di Lama di Reno potrebbe, infatti, creare rilevanti problemi occupazionali e comprometterebbe il futuro di un insediamento produttivo di tradizioni storiche nella montagna e nella Provincia bolognese.

di un protocollo d'intesa tra azienda, RSU, organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, istituzioni locali, Regione Emilia Romagna, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e Ministero Con tale protocollo tutte le parti si assumono l'impegno di sostenere la ricerca da parte dell'azienda di eventuali acquirenti disponibili a proseguire l'attività di produzione della carta nello stesso stabilimento di Lama di Reno. A questo scopo, sia i Ministeri competenti che le istituzioni locali sono impegnati a realizzare il progetto «La filiera delle cartiere», presentato dal tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'ambiente. Esso prevede il miglioramento della fornitura delle materie prime per la produzione di carta riciclata, la ricerca di uno sbocco più certo di mercato in linea con le disposizioni concernenti gli «approvvigionamenti verdi» della pubblica amministrazione, la riduzione del costo dell'energia attraverso una maggiore efficienza degli impianti e un notevole utilizzo degli scarti di produzione cartaria. In alternativa, il protocollo prevede la possibilità da parte del gruppo di cedere lo stabilimento anche per altre iniziative produttive, finalizzate alla reindustrializzazione dell'area e al mantenimento dei livelli occupazionali. L'impegno assunto dall'azienda con il protocollo prevede un termine al 31 dicembre 2007, data in cui essa si riterrà libera da ogni vincolo. Per questa ragione, il protocollo prevedeva che il Governo supportasse la domanda rivolta al Ministero del lavoro della cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività della durata di 12 mesi. A tutt'oggi, il Ministero del lavoro ha concesso la cassa integrazione solo fino al mese di giugno, mentre per il suo prolungamento fino alla fine del 2007 è necessaria la concessione della cassa integrazione in deroga, prevista per casi di particolare gravità, per la quale si è in attesa dell'emanazione del relativo decreto attuativo da parte delle amministrazioni competenti. Il Governo, quindi, si dichiara intenzionato ad attuare scrupolosamente tutti gli impegni contenuti nel protocollo d'intesa, il quale prevede, peraltro, una prima verifica entro aprile 2007, in modo che sia garantita, come richiesto dagli interroganti, una prospettiva positiva per lo stabilimento di Lama di Reno, per quel comparto produttivo e per i lavoratori interessati.

Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Bubbico per la risposta all'interrogazione che ritengo pienamente soddisfacente. Il Sottosegretario ha infatti dichiarato, in modo molto puntuale, l'impegno del Governo ad attuare in modo scrupoloso - così ha detto ‑ il protocollo d'intesa tra le diverse parti, sottoscritto presso il Ministero dello sviluppo economico il 13 dicembre scorso. In modo particolare si è riferito al problema della cassa integrazione, poiché, come egli ha detto, è necessario giungere con questo strumento fino alla fine dell'anno in corso per consentire la ricerca di altri soggetti imprenditoriali in grado di continuare l'attività produttiva dello stabilimento di Lama di Reno. Poiché il Ministero del lavoro ha concesso solo la cassa integrazione straordinaria fino al giugno di quest'anno, è per l'appunto necessario, come il Sottosegretario ha detto, operare affinché sia concessa la cassa integrazione in deroga fino alla fine del 2007. Mi pare che questo sia un impegno assunto dal Governo e per questo sono molto soddisfatto della risposta, come pure sono soddisfatto perché è stata ribadita la volontà di sviluppare il progetto cosiddetto della filiera delle cartiere, in considerazione del fatto che nella Valle del Reno, vicino a Bologna, vi sono numerosi stabilimenti di questo genere, anche se ovviamente non è solo un problema bolognese. Questo andrà nella direzione di favorire tutti gli impianti che producono carta riciclata, penso sia necessario creare un mercato per questi stabilimenti (ovviamente non solo per quello bolognese) attraverso politiche pubbliche forti, capaci di incentivare il riciclaggio della carta e quindi anche la sostenibilità ambientale della nostra economia. Ringrazio ancora il Ministro e naturalmente sono disponibile, insieme con altri parlamentari della mia città, a collaborare con il Ministero al fine di ottenere il risultato voluto e cioè la salvezza di quell'importante stabilimento.